la parola a lei, senatore Cossiga. COSSIGA *(Misto)*. Signor Presidente, signori senatori, credo mio dovere motivare in quest'Aula le mie dimissioni dal Senato, Camera augusta del Parlamento nazionale che è in democrazia il solo "sovrano legale" nella Repubblica, Parlamento nazionale al quale mi onoro di essere stato eletto ormai quasi cinquant'anni fa, e di averne fatto parte, spero non indegnamente, per quasi lo stesso periodo, se non si tiene conto della mia quasi del tutto occasionale presenza al Quirinale. Questo dovere è reso più forte dall'avere anche presieduto questa Assemblea. Dopo aver pronunziato queste mie, spero non troppo tediose parole, lascerò doverosamente l'Aula, per assicurare ai membri del Senato, con la mia non presenza, maggiore libertà di parola e serenità di giudizio. Non ho rassegnato le dimissioni perché, come è mio convincimento, sarebbe ormai necessario e opportuno sopprimere l'istituto del senatore a vita o modificarlo in coerenza con il carattere elettivo della rappresentanza democratica, o anche riformarlo, riconoscendo ai senatori a vita tutti i diritti, le facoltà e le prerogative dei senatori elettivi, salvo il diritto di voto, per non interferire nei risultati del voto del popolo, che in democrazia è l'unico "sovrano reale". Questo sarà un problema che il Parlamento affronterà e sul quale adotterà le sue decisioni. Io mi sono assunto le mie responsabilità, e quando ho ritenuto che una rovinosa crisi politica potesse verificarsi con inevitabili nuove elezioni effettuate con questo sistema elettorale e nella situazione di complessa incertezza che domina entrambe le coalizioni, ho votato anche la fiducia al Governo di centrosinistra, pur non facendo parte della maggioranza, e anche i suoi più importanti provvedimenti quali la legge finanziaria e la legge di bilancio, non stando certo a me modificare la Costituzione e non ritenendo di dovermi, per così dire, degradare rispetto agli altri senatori a vita, dato che la mia isolata proposta formulata ad essi, ancor prima delle elezioni, quando già ad una semplice lettura della nuova legge si delineava la difficoltà di costituire una maggioranza al Senato, di astenerci dal voto qualora esso determinasse maggioranze non esistenti o in contrasto con i risultati del voto popolare, non ha avuto favorevole esito. Mi sono dimesso per tutelare le prerogative del Parlamento connesse alla sua antica ed essenziale funzione di controllo sull'Esecutivo, esercitata con gli istituti dell'interpellanza e dell'interrogazione, istituti da considerarsi quasi quasi superati e ormai desueti, se devo giudicare dal numero delle interpellanze e delle interrogazioni, ma ve ne faccio grazia, da me rivolte al Governo e ai singoli Ministri a cui, nonostante i solleciti della Presidenza, che ringrazio, mai è stata data risposta! Mi sono dimesso per tutelare il Senato e l'offesa a me in quanto suo membro recata, quando, invero assente il cortese Ministro dell'interno dal nostro Paese, un ufficio del suo Ministero, ed in sostituzione alla risposta...

ha ritenuto di rispondere ad una mia interpellanza con una dichiarazione resa alla stampa da un suo funzionario. In vero, trasformata per cortesia e per consiglio prudente e gentile della Presidenza, in interrogazione a risposta scritta, il Ministro dell'interno ha con gentilezza risposto per iscritto, negando che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza avesse dato denaro a dei giornalisti, e per negare che, a suo giudizio, questo non era forse mai avvenuto o ancora avvenisse, non praticandosi quindi, a suo avviso, più questa, diciamo così, nota prassi d'origine giolittiana! Egli mi ha risposto, ripeto, con assoluta gentilezza e credo che egli, per quel che sa, abbia certamente detto la verità. Sino a ieri non mi era stata data risposta dal Ministro dell'interno all'interpellanza, poi trasformata in interrogazione a risposta scritta, con la quale chiedevo chiarimenti in ordine all'attività del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle DIGOS di Milano e di Roma in merito all'inchiesta della procura della Repubblica di Milano sulla "*extraordinary* *rendition*" operata da agenti della CIA nei confronti di un cittadino egiziano. Soltanto ieri, appunto, il Ministro dell'interno ha risposto alla mia interrogazione. A motivo del contenuto della risposta del Ministro ritengo mio dovere politico e morale chiedere pubblicamente e formalmente scusa al prefetto Gianni De Gennaro per le dure critiche e accuse da me più volte rivoltegli in quest'Aula e fuori di quest'Aula. Il Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto De Gennaro, si è comportato con assoluta lealtà nei confronti del Governo, fornendogli in relazione al caso SISMI tutte le informazioni che egli aveva acquisito; e debbo altresì riconoscere che con grande spirito di collaborazione istituzionale con il Governo, prima e durante le indagini che hanno coinvolto agenti del SISMI, si sono comportati i magistrati del pubblico ministero della procura della Repubblica di Milano. Altro appartiene alla responsabilità politica del Governo. Intatta rimane la mia stima e il mio affetto per il generale Nicolò Pollari, tuttora perseguitato da un'assurda inchiesta giudiziaria che già tanto nocumento ha arrecato al nostro apparato di sicurezza e alle nostre relazioni, anche nel campo della lotta al terrorismo, con una grande Nazione alleata e amica. Legato ad un mondo ormai tramontato, nel quale la sinistra era la sinistra, la destra era la destra e il centro era il centro, la sinistra e il centro d'ispirazione sociale democratica cristiana e socialista erano a favore dell'intervento pubblico nell'economia, per un'industria e un sistema bancario di Stato, per un mercato controllato e guidato dai pubblici poteri, e la destra e il centro d'ispirazione liberale erano a favore dell'economia di mercato, delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, tutte aborrite dalla sinistra socialista e dal centro d'ispirazione democratica cristiana, mi oriento a disagio e poco comprendo nell'attuale situazione ideologica e politica sia per quanto riguarda il centro-destra sia per quanto riguarda il centro-sinistra. Per questi motivi, oltre che per la ingravescente età che sempre più mi rende mentalmente e fisicamente non idoneo ad esercitare con la dovuta assiduità e diligenza le delicate e complesse funzioni di membro di questa Alta Camera del Parlamento nazionale, ho rassegnato le dimissioni da senatore della Repubblica. Spetta ora a voi, signori senatori, valutare le mie motivazioni e decidere sulle mie dimissioni.

Al Gruppo Misto sono riservati complessivamente 15 minuti. I senatori a vita che intendono intervenire avranno a propria disposizione un autonomo tempo di dieci minuti ciascuno; ai senatori che dissentono dal proprio Gruppo sono attribuiti complessivamente 15 minuti.

non credo di aver capito male, ma stamattina il Presidente di turno ha dichiarato che avremmo continuato nel pomeriggio le votazioni sul decreto-legge n. 299; adesso vedo che c'è un cambiamento.

Presidente, stavo cercando di spiegare al Segretario generale una questione un po' particolare. La dichiarazione di voto per il Gruppo UDC la farà il collega Buttiglione perché io ritengo che non si debba votare e quindi non è che sono in dissenso dal Gruppo:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Cossiga rappresenta una delle figure più importanti nella storia recente della Repubblica e ha svolto un'opera di fondamentale importanza anche nella fase di transizione tra la cosiddetta Prima Repubblica e la cosiddetta Seconda Repubblica. Successivamente, la sua posizione politica è stata sempre quella di chi pungolava, ricordando come tale transizione non sia in effetti avvenuta come la Prima Repubblica venga sempre più rimpianta quanto più si mostra l'incapacità del nuovo ceto politico di costruire le condizioni della Seconda Repubblica. Qualunque cosa si pensi delle sue posizioni politiche, egli ha sempre avuto grande onestà e generosità personale, con la quale ha condotto le sue battaglie e ci ha resi attenti alle incongruenze, alle contraddizioni e ai limiti del sistema che siamo venuti costruendo a pezzi e a bocconi, senza - temo una precisa linea guida direttrice e senza una visione architettonica complessiva. Capisco le ragioni di amarezza personale che lo inducono a dare queste dimissioni mi stupisco che le questioni da lui sollevate abbiano trovato così poca eco. Immagino che sarebbe giusto, in questo momento, domandarci quale sia l'atteggiamento corretto che è necessario tenere in un Paese democratico, ma impegnato nella guerra al terrorismo su vicende come quelle che hanno recentemente sconvolto i nostri Servizi segreti. Credo che molte cose che egli sostiene riguardo al carattere un po' operettistico di servizi segreti che sono spiati e le cui telefonate sono intercettate dalla magistratura, dovrebbero farci riflettere. Vedo invece che un dibattito al riguardo stenta a decollare

se l'Italia ritenga di essere parte, insieme con tutta l'Unione Europea, di una comunità atlantica che difende la libertà del mondo o se invece riteniamo che gli Stati Uniti siano una potenza imperialistica contro la quale è lecito e giusto che i popoli del mondo si ribellino. Queste grandi questione politiche, che stanno dietro la richiesta di dimissioni, credo che non troveranno molta eco nel dibattito in quest'Aula. Noi invece riteniamo che si tratti di questioni politiche fondamentali ed apprezziamo il modo con cui il presidente Cossiga ha tentato di porle. Questo è uno dei motivi per i quali riteniamo che le dimissioni vadano respinte. Al di là di questo giudizio in particolare, rimane la stima verso una persona la quale nobilita con passione, decisione e coraggio un dibattito politico che di passione, di coraggio, di spirito di sacrificio, di volontà di cercare la verità senza compromessi ha sicuramente bisogno. Ovviamente, nel nostro Gruppo vige la libertà di coscienza su questi temi, ma credo che la grande maggioranza dei suoi membri si atterrà all'indicazione di votare per respingere le dimissioni del senatore Cossiga.

questa sia una discussione importante, che non riguarda esclusivamente un collega senatore, pur così autorevole come il presidente Cossiga. Penso, tra l'altro, che chi ama la politica intesa come conflitto, ma anche come raffinata costruzione istituzionale e quindi chi detesta l'antipolitica, il populismo, il plebeismo, nell'articolata accezione gramsciana, non può che desiderare che il presidente Cossiga sia fra noi su questi banchi, caleidoscopio di tutte le contraddizioni, le ambivalenze e anche le anomie della politica, nella quale la provocazione è sempre portata sino al limite della rottura e il paradosso, coltivato spesso con sapiente accortezza, cela sempre allusioni a verità più o meno nascoste. Il presidente Cossiga, certo, è uomo della Prima Repubblica, ma la Seconda Repubblica, a mio avviso, è naufragata nella tenaglia della fuga dalla democrazia, che è nelle viscere della globalizzazione liberista; la terza Repubblica dovremo e potremo ancora cominciare a costruirla insieme, ripartendo dalle grandi narrazioni di massa. Sia concesso ad un anziano dirigente politico come me - e me ne scuso con le compagne e i compagni più giovani anche del mio Gruppo - un ricordo personale, un piccolo ma modesto segmento del vissuto di tempi aspri e convulsi. Nel 1987 - ero allora segretario di Democrazia Proletaria - ho formalmente denunziato, in base all'articolo 90 della Costituzione, l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga... PRESIDENTE. Senatori Viceconte e Storace, vi invito

dopo che, con provocatoria rivendicazione, aveva rivelato di aver conosciuto, costruito e collaborato a «Gladio», che io ritenevo e ritengo essere stata un'incostituzionale associazione sovversiva dell'ordinamento repubblicano e non un'associazione di patrioti, come egli sostiene. Il presidente Cossiga in quell'occasione mi chiamò: discutemmo più e più volte, bisticciammo aspramente, ma iniziò allora un dialogo che non si è poi mai interrotto. Io continuo a ritenere che Cossiga sia un cattolico stalinista; egli ritiene - com'è solito dire - che io sia un illuso, come tutti i comunisti libertari. Mi posso quindi permettere ora di chiedere al presidente Cossiga, anche a nome dell'intero Gruppo, di non interrompere il dialogo, anche sui banchi del Senato, i quali sarebbero meno attraenti e interessanti senza di lui.

Il presidente Marini, intendendo così anche il precedente della scorsa legislatura, ha interpretato il dibattito in seno all'Assemblea costituente, e in particolare l'intervento di Umberto Terracini, come ammissibilità delle dimissioni dei senatori nominati a vita, nella considerazione che nessuno può essere costretto a mantenere un pubblico ufficio contro la propria volontà. Non è l'unica interpretazione che può essere addotta sul piano costituzionale: legittimamente si può ritenere, in questa complessa materia, che altre debbano essere le interpretazioni. Comunque, non è di questo che ci parlano le dimissioni del presidente Cossiga; non è questo il punto centrale. Queste, invece, ci parlano - voglio sottolinearlo - di un punto fondamentale, primario nelle sue motivazioni or ora addotte: delle prerogative del Parlamento e della sua centralità nel rapporto con il Governo soprattutto per quanto concerne il potere, anzi, il diritto-dovere di ogni parlamentare di esercitare il sindacato ispettivo con interpellanze, interrogazioni, mozioni nei confronti di atti commessi o anche di omissioni dell'Esecutivo. È di questo che ci parla il presidente Cossiga. Io non entro nel merito delle questioni poste, su cui le opinioni possono coincidere o meno; anzi, per non essere ipocrita, dico che sui due temi specifici citati dal presidente Cossiga, nel merito (cioè per quanto riguarda l'inchiesta della procura della Repubblica di Milano sulle

il sottolineare, da parte del presidente Cossiga (e su questo sono d'accordo), la straordinaria attenzione, cura per le prerogative del Parlamento, per la sua centralità anche nei confronti dell'Esecutivo;

nelle materie non previste dalla Costituzione. Io credo che questo tema, a cui alludono le dimissioni del presidente Cossiga, debba stare a cuore ad ogni parlamentare che ritiene sia centrale nella nostra Costituzione, come ha detto il *referendum* di giugno, il Parlamento.

svolgere poche considerazioni per invitare l'Aula a respingere le dimissioni del presidente Cossiga

quanto ci ha offerto in esame il presidente Cossiga, perché ritengo che lui sieda in quest'Aula in virtù di una previsione costituzionale che credo il legislatore, all'epoca, abbia previsto per dotare questa Camera

di voto concessa ai senatori a vita. A mio avviso, tale istituto dovrebbe rimanere così com'è previsto dalla Costituzione, così come *de iure* *condito* noi lo abbiamo applicato e continuiamo ad applicarlo. In verità, il presidente Cossiga già in altre epoche ci ha insegnato che picconando probabilmente riusciva a smuovere equilibri e a crearne di nuovi. Ritengo che questa sia un'ulteriore picconata da parte sua al nostro assetto costituzionale, forse cercando di farci intendere che è necessario rivedere tale istituto: forse il presidente Cossiga lo fa a modo suo, appunto picconando e sottoponendo all'attenzione dell'odierno legislatore la necessità di rivedere un istituto che, dal suo punto di vista, non è più attuale.

le ragioni che hanno indotto il presidente Cossiga a rassegnare le dimissioni dal Senato, al di là del caso specifico che le ha determinate, credo meritino una particolare attenzione. soprattutto, a quella parte della lettera in cui il presidente Cossiga afferma che l'istituto dei senatori a vita, di diritto o di nomina presidenziale, è del tutto anacronistico in una democrazia rappresentativa e che le sue dimissioni sono un atto di coerenza politica, istituzionale e morale, aggiungendo di ritenere il Parlamento - come ha ripetuto anche prima - l'unico e supremo «sovrano legale» del nostro Stato democratico, perché rappresentativo per libero mandato elettorale dell'unico «sovrano reale» nello Stato stesso, cioè il popolo. Come si vede, la lettera del presidente Cossiga è particolarmente centrata su alcuni punti irrinunciabili e fondamentali della nostra Costituzione: il Parlamento come sovrano legale, il popolo come sovrano reale, il rispetto assoluto della volontà popolare, la presenza e il ruolo dei senatori a vita. La domanda che dobbiamo porci è se in Senato vi è stato il rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, laddove afferma che la sovranità appartiene al popolo. La risposta che noi diamo è negativa. La volontà popolare é stata ripetutamente manomessa dal voto dei senatori a vita che, sebbene non eletti, ma soltanto nominati, hanno consentito con il loro voto determinante, in occasione dell'esame della legge finanziaria, di salvare il Governo Prodi. Un Governo che ha incassato la fiducia di metà dei senatori eletti contro un'altra metà del Senato e che, per sopravvivere, ha dovuto ricorrere al voto determinante di chi, perché nominato, non rappresenta la volontà popolare. Una forte contraddizione, quindi, tra le affermazioni di principio e i comportamenti reali ha contraddistinto la presenza in Senato dei senatori di diritto e di nomina presidenziale; una presenza che ha indubbiamente manomesso le regole democratiche e ha aggravato ulteriormente la condizione politica in cui versa il Paese. Una condizione politica che vede il Governo ancora non pienamente legittimato per l'incertezza dell'esito elettorale, per la superiorità dei consensi ottenuti dal Polo al Senato, per l'esigua differenza di voti che ha determinato il risultato della Camera e per gli inevitabili e per gli inevitabili errori di calcolo legati al conteggio di milioni di voti. Ciononostante vi è stata una forzatura inaccettabile, con la sottomissione dei senatori a vita ad un disegno non rispettoso delle regole democratiche, che rende inutile addirittura la consultazione elettorale, che alimenta le divisioni, i conflitti e la sfiducia dei cittadini nei confronti delle nostre istituzioni.

la più alta carica dello Stato, vi era almeno uno sforzo complessivo di apparire garanti dell'unità nazionale, di stare al di sopra e al di fuori di ogni posizione politica. Oggi, invece, non si ha alcuna remora a mettersi al servizio, tra l'altro in modo acritico e strumentale, di una parte politica per combattere un'altra parte politica. Tutto ciò credo getti un'ombra sulla presunta imparzialità che avrebbe caratterizzato il loro settennato. Infatti, domando: che significato possiamo dare oggi al messaggio inviato da Ciampi alle Camere sul pluralismo dell'informazione radiotelevisiva? Nasceva questa esigenza dalla necessità di garantire democrazia e libertà in un settore così delicato come l'informazione o nasceva dall'esigenza di dare una mano alle opposizioni di centro-sinistra? Che significato possiamo poi dare al decreto con il quale l'allora presidente Scalfaro sciolse le Camere a seguito delle dimissioni dell'allora presidente del Consiglio Ciampi? Nasceva forse dall'esigenza di dare vita ad un nuovo Parlamento sulla base di una nuova legge elettorale o nasceva piuttosto dalla volontà di consegnare il Paese alla gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto? Quale significato possiamo noi dare, poi, all'iniziativa di Scalfaro, quando, a seguito delle dimissioni di Prodi, favorì la nascita del Governo D'Alema con una maggioranza parlamentare dove vi erano i voti determinanti di parlamentari usciti dal Polo delle Libertà? Nasceva anche questa dall'esigenza di dare vita ad un nuovo Governo o dall'esigenza di impedire nuove elezioni politiche come veniva richiesto dall'opposizione?

Che dire poi del comportamento dei senatori non eletti, ma nominati per avere illustrato la Patria, e che oggi brillano esclusivamente per illustrare le gesta del Governo Prodi. Che senso ha la loro pervicacia, la loro supponenza e la loro arroganza verso la democrazia, quando proprio perché hanno rappresentato la Patria dovrebbero continuare a rappresentarla nella sua interezza, nel rispetto del responso elettorale, evitando di alimentare lo scontro e la sopraffazione? Quale giudizio dovremmo esprimere verso quei senatori a vita che siedono in Senato solo ed esclusivamente un attimo prima di votare la fiducia a Prodi per poi, immediatamente dopo, abbandonare l'Aula? Quando mai il prestigio e l'autorevolezza delle più alte cariche sono stati messi in queste condizioni? Avremmo preferito non aprire una polemica di queste dimensioni nei confronti di chi dovrebbe continuare a rimanere al di sopra e al di fuori di ogni contrapposizione politica. La nobiltà e l'altezza delle cariche ricoperte doveva metterli al riparo dalle polemiche della battaglia politica quotidiana. Purtroppo si è preferito scegliere la strada della contrapposizione e dello scontro e ciò ha reso inevitabile considerarli come un vero e proprio partito politico, collocato rigidamente a sinistra, a fianco anche di quella sinistra legata ai gruppi più radicali e più antisistema. Coloro che hanno rappresentato le più alte cariche sono entrati nella vicenda politica a gamba tesa e, pur essendone consapevoli, si sono spogliati di quella autorevolezza che doveva contraddistinguere la loro presenza nel Senato della Repubblica. Se le cose dovessero continuare come sono avvenute fino ad oggi è evidente che dovremmo aprire una questione davanti al Paese, in termini più marcati e più incisivi, per rappresentare una grave anomalia presente nel nostro sistema democratico a causa del voto usato dai senatori a vita come grimaldello per manomettere e sovvertire le regole della nostra democrazia. Noi continuiamo comunque a sperare che si torni quanto prima a percorrere la strada maestra del rispetto della volontà popolare e continuiamo a sperare che prevalga il senso dello Stato, le ragioni del Paese, la soluzione dei problemi reali. Le condizioni di paralisi delle Camere, soprattutto quella del Senato, la insicurezza determinata dalla instabilità politica, la mancanza di una governabilità vera dovrebbero indurre anche i senatori a vita a favorire punti di incontro fra i due poli per trovare soluzioni innovative, che superino anche l'attuale quadro politico. Nella coalizione di Governo vi sono sintomi di grande insoddisfazione e di legge insofferenza; vi è la sensazione di vivere di vivere in un recinto che non lascia spazio e respiro ad una vera politica di riforme; vi è ormai la consapevolezza di una condizione asfittica che spegne ogni slancio di novità ed ogni speranza di cambiamento. Occorre quindi superare le barriere per incontrarci su un terreno diverso, più alto e più nobile, dove siano possibili convergenze più ampie e politiche più avanzate. Il presidente della Repubblica Napolitano ha invitato i poli ad aprirsi al confronto e al dialogo, ma anche alla collaborazione sulle grandi emergenze nazionali. Noi abbiamo accolto questo invito. Aspettiamo che altri facciano È auspicabile che anche il presidente Cossiga, che invitiamo chiaramente a rimanere sui banchi del Senato, e gli altri senatori a vita siano in grado, più di altri, di accogliere tale invito e di assecondare le nuove aspirazioni che nascono dal Parlamento e dal Paese.

sia mio dovere intervenire. Qui c'è un problema di principio e un problema che vorrei definire di fatto. Se attraverso le debite forme sarà soppresso l'istituto dei senatori a vita, purché si dia il tempo di potersi ripresentare agli elettori, come ho fatto per 45 anni, non non potrei certamente sollevare obiezioni. Vorrei però non si confondessero questi temi. La Costituente fece una scelta motivata, anzi vorrei ricordare che, per dare una certa continuità alla prima legislatura, la Costituente stessa creò, per la prima legislatura, la figura dei senatori di diritto,

18 aprile, forse qualcuno lo ricorda, dette ai partiti di centro una notevole maggioranza assoluta, ma mai nel corso della legislatura vi fu una votazione nella quale si andò contro quello che era stato il responso popolare. Questa è storia passata e può avere o meno importanza. Per il resto, la sensibilità personale dell'onorevole Cossiga è tutta particolare. Ricordiamo le dimissioni che rassegnò da Ministro dell'interno e certamente non aveva responsabilità lui se, dolorosamente, lo Stato venne sconfitto e Moro fu ucciso e non si venne a capo di quella terribile congiuntura di carattere nazionale. Io vorrei veramente invitare l'onorevole Cossiga

aspetto, nessuno deve temere una forma di utilizzo delle nostre possibilità di voto per forzare delle situazioni. Noi rispondiamo prima di tutto alla nostra coscienza quando votiamo, non abbiamo dei calcoli prefabbricati o delle finalità di carattere indiretto. In una delle ultime votazioni sono trovato in difficoltà, perché gli emendamenti precedenti erano passati per un solo voto: trovandomi dinanzi al problema dei due ruoli della magistratura,

ad un ruolo. Quindi, mi trovavo, con il mio voto, a dover stabilire i due ruoli della magistratura: in quel caso mi sono seduto e non ho partecipato al voto. Credo di aver fatto il mio dovere. il mio dovere. Ritengo che lavorando intensamente, con molta umiltà e con molta passione, per questa gloriosa istituzione parlamentare, noi non dobbiamo chiedere scusa a nessuno né dobbiamo fare dei cambiamenti.

è stato una delle persone più importanti della Prima Repubblica. Voglio sperare che il dibattito non si incentri su motivazioni di ordine ideologico, perché io ho un percorso diverso dal collega Buttiglione, anche se io e lui - ne sono onorato

ha lavorato, ma non posso affrontare le dimissioni del senatore Cossiga in funzione della Prima Repubblica, quando vigeva un Governo *ad* *excludendum* verso alcune forze politiche, ad una delle quali mi onoro di aver fatto parte.

la risposta del ministro Amato in una sceneggiata. È una cosa seria ciò che il collega Cossiga ha scritto nella sua lettera di dimissioni. Prendiamo atto che ha chiesto scusa

rinviare la votazione sulle dimissioni del senatore Cossiga e chiedere al Ministro dell'interno di venire qui e acclarare ciò che ha scritto in risposta, sotto forma privata, al senatore Cossiga? Perché non venire qui?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dimissioni del senatore Cossiga pongono l'accento su una questione di rilevanza costituzionale, ossia il ruolo rivestito nell'attività parlamentare dei senatori a vita. Noi respingeremo decisamente la richiesta di dimissioni del senatore Cossiga, Presidente e, come molti hanno ricordato, uomo della Prima e della Seconda Repubblica che deve continuare a fornire la sua importante esperienza al servizio del Parlamento e, quindi, del Paese. L'esperienza e la saggezza sono qualità necessarie delle quali noi,

di una condizione che si è creata dopo sessant'anni. Ebbene, è giusto che la saggezza e l'esperienza possano intervenire di volta in volta sia a favore del centro-destra sia a favore del centro‑sinistra, perché questo sta accadendo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo respingerà la richiesta di dimissioni del presidente Cossiga e non lo farà né per ragioni di cortesia, né per ragioni giuridiche, anche se interessante è la prospettazione che il presidente D'Onofrio ci ha già proposto in quest'Aula in un'occasione precedente e anche se convengo con quanto il presidente Andreotti ci ha voluto oggi comunicare. Lo faccio per ragioni politiche di natura generale, colleghi, e per ragioni istituzionali, giacché l'aggettivo "generale" credo sia adatto a definire l'attività politica e istituzionale di un uomo che si definisce non di parte e che tale io credo possa essere riconosciuto da ciascuno di noi. E lo faccio prendendo spunto dall'ultima parte dell'intervento del presidente Cossiga, una parte che mi ha molto colpito. Lo faccio innanzitutto rallegrandomi per l'esito della vicenda che lo ha contrapposto al ministro Amato e rallegrandomi per il fatto che, anche per il tramite di questa vicenda, un interrogazione a risposta scritta, il presidente Cossiga, ha avuto piena soddisfazione, garanzia questa che credo tocchi e sia cara a ciascuno di noi. Ma lo faccio - dicevo - con riguardo all'ultima parte dell'intervento odierno del presidente Cossiga, una parte in cui egli fa riferimento ad un suoproprio smarrimento, uno smarrimento politico, quello derivante dall'essere legato ad un mondo ormai tramontato - dice - nel quale le stesse posizioni della sinistra, del centro e della destra si confondono e non rispettano più quelli che erano i binari consueti della politologia classica; uno smarrimento che ci richiama probabilmente alle parole di un altro grande senatore a vita, Eugenio Montale, che descrive l'ultima parte della sua vita come parte nella quale la bussola va girando all'impazzata e il calcolo dei dadi più non torna. Questo smarrimento, colleghi, se vogliamo guardare con schiettezza dentro di noi a questo passaggio del nostro Paese, credo che tocchi tutti e sia conosciuto da ciascuno di noi che ha subito anche nelle forze politiche di appartenenza profonde trasformazioni; penso alla sua vicenda politica e a quella del suo partito, presidente Matteoli, e penso a quella del mio partito o a quella del partito della Margherita. Penso sia uno smarrimento che in qualche modo, per quanto possiamo dissimularlo e fingere che non esista, ci prende di fronte alla modernità, al tempo nuovo, ai nuovi problemi, ai nuovi doveri, alle nuove responsabilità e alle nuove domande alle quali la politica è chiamata. Penso che ciascuno di noi in momenti come questo senta più saldamente la necessità di ancorarsi a ciò che ha di più consueto e caro: certo, le radici ideali delle nostre forze politiche di appartenenza, ma forse, soprattutto per noi che sediamo in Aula, la fedeltà alla Costituzione e l'affezione alle istituzioni. Quando i Costituenti previdero che gli ex Presidenti della Repubblica sedessero di diritto al Senato a questo pensavano, al fatto cioè che comunque ci fosse un presidio forse più ancorato, per esperienza, per tradizione,

alle istituzioni. Questa è la ragione per cui il presidente Cossiga, il presidente Ciampi, il presidente Scalfaro siedono qui e spesso - lo confessiamo - ci rammentano questa fedeltà e questo quadro, anche nei momenti in cui più aspro è qui il confronto tra di noi; non una carica onorifica, quindi. Mi scusi, senatore Baldini, ma non condivido le sue argomentazioni. Rileggo il dibattito alla Costituente e trovo che la presenza degli ex Presidenti della Repubblica al al Senato garantisce la piena e libera esplicazione della sovranità del Parlamento. Sarebbe paradossale che a loro fossero riconosciuti per questa ragione diritti diminuiti. diminuiti. Nell'ultima parte dell'intervento del presidente Cossiga si coglie un tratto, che apprezziamo, quello di ritenersi forse troppo vecchio e troppo stanco; diciamolo con parole più colloquiali rispetto a quelle che lui ha usato. Su questo aspetto le devo pur dire che lei non è credibile perché chi con lei ha sempre polemizzato, ma ha anche convenuto sempre o qualche volta, non può comunque rintracciare nei suoi atteggiamenti mai l'ovvio, mai la pedissequa ripetizione di un punto di vista, dello stesso punto di vista né sul mondo, né sul Paese, né sulle politiche, né su tante altre questioni. Lei non è mai stato uguale a se stesso nel proporre il suo punto di vista del mondo. Penso che anche questo serva al Senato. È per tutte queste ragioni che il mio Gruppo convintamente

Personalmente sono anche poco convinto della legittimità di quello che stiamo per affrontare e ritengo che le dimissioni di un senatore di diritto e a vita non siano nella disponibilità neppure dell'interessato, salvo

che ci dice che furono già votate delle dimissioni, ma se un errore rischia di creare una prassi, il proseguire su questo errore rischia di far diventare diabolico il Senato. Comunque sia, dovendo esprimere un voto, proprio per la stima e la simpatia che ho per il presidente Cossiga, il mio voto sarà a favore delle sue dimissioni in quanto è lui ad averle chieste. E se devo rispettare la sua volontà e devo ascoltare le motivazioni che lui stesso ha portato nell'intervento di quest'oggi reso all'Assemblea, non posso che rispettare la sua volontà e le sue motivazioni con un voto positivo alle sue dimissioni. E lo dico francamente contro il mio interesse perché sono convinto che, semmai dovessero essere approvate delle dimissioni, non so neppure se domani non ci troveremmo comunque ancora senatore il presidente Cossiga. Ma se queste dimissioni non vorrei che ciò spingesse il Presidente della Repubblica alla nomina di un ulteriore senatore a vita, che sicuramente andrebbe a sedersi nell'altra parte in maniera più convinta di quanto abbia fatto fino a d'oggi l'amico e collega

Signor Presidente, durante il presente dibattito si è fatto riferimento, ancora una volta, ad alcune mie decisioni e al mio operato come Presidente della Repubblica. quindi intervenire per riaffermare che come Presidente della Repubblica la mia linea di condotta è stata sempre quella di rispettare e di far sì che in ogni provvedimento al mio esame fosse rispettata la Costituzione, nei suoi princìpi e nelle sue norme. Non ho mai ceduto a pressioni di maggioranza o di opposizione, né a sollecitazioni di altra natura. Come senatore a vita ho e continuerò ad avere come miei riferimenti la Costituzione e la mia coscienza eserciterò, secondo l'una e l'altra, i miei diritti di componente di questa Assemblea. Per quanto riguarda le dimissioni del senatore Cossiga, per i motivi che sono stati illustrati anche dal senatore Andreotti, voterò per respingerle. *(Vivi

non ho dubbi circa la legittimità e l'efficacia del ruolo degli ex Presidenti della Repubblica e dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. Non ho dubbi sulla legittimità del loro ruolo e sull'efficacia della loro presenza in questa nostra Aula e rispetto ai problemi e alle esigenze del nostro Paese. Condivido a questo riguardo quanto ha detto l'onorevole Andreotti e ora ha ribadito il presidente Ciampi. Desidero semplicemente soggiungere un aspetto più propriamente politico. Seggo in Parlamento da 35 anni; ho vissuto tante battaglie politiche e durante queste lunghe e importanti vicende della mia vita, che hanno coinciso con gran parte della vita della nostra Repubblica, ho dovuto spesso contrastare, anche duramente, le scelte politiche o i comportamenti di Francesco Cossiga, e ho avuto modo di condividere sue scelte e di sostenere sue decisioni in momenti cruciali per la vita della Repubblica italiana. È anche per tutto questo che io ritengo che la presenza di Francesco Cossiga, la permanenza del senatore Cossiga nella nostra Aula sia motivo di validità, di forza, di efficacia, un contributo importante al quale il Senato non deve rinunziare, e per questo invito il Senato a respingere le sue dimissioni, e così io mi comporterò. Presidente, io non volevo intervenire, perché, essendo un voto segreto,

i rappresentanti seduti ai banchi del Governo tributino una vera e propria *standing ovation...

del tutto legittimamente, la permanenza del senatore Cossiga in quest'Aula. Io, però, credo che questo voto non debba essere soltanto inteso come un voto di cortesia che si suole, e in questo caso forse si deve, tributare ad un personaggio della levatura politica del senatore Cossiga, credo che non debba sfuggire che esso assume obbligatoriamente un significato politico ben preciso, perché il senatore Cossiga si dimette anche in seguito a fatti ben precisi. L'abbiamo sentito con le nostre orecchie, in quest'Aula, proferire parole estremamente gravi anche nei confronti del Capo della Polizia - e questo non può sfuggire - su una vicenda che coinvolge l'attività ed il buon nome internazionale dell'Italia, che comunque è sempre la vicenda Abu Omar, sulla quale continuerò ad intervenire finché non sarà chiarita del tutto, che invece si complica sempre di più. L'abbiamo visto anche stamattina sui giornali: c'è la questione del pubblico ministero Spataro, che interviene duramente contro una parte del disegno di legge

con l'apporto fondamentale della maggioranza, respingerà le dimissioni del senatore Cossiga, conseguentemente ed inevitabilmente vorrà dire che in qualche modo vengono sposate le tesi del senatore Cossiga che su questo tema, tra l'altro, io condivido pienamente. E allora si aprirebbe, si deve aprire immediatamente e susseguentemente, un esame parlamentare sulla questione di come si sia comportata la procura di Milano sulla vicenda Abu Ornar,

di come possono operare i nostri Servizi, di quale sia il rapporto tra il Parlamento e la magistratura; e, guarda caso, ogni volta viene fuori la questione della procura di Milano. Se non affronteremo e risolveremo una volta per tutte questo problema, saremo sempre un Parlamento e un Governo a sovranità limitata perché c'è una procura i cui magistrati in alcuni casi si trovano *legibus soluti* e agiscono in qualsiasi modo. Perché il senatore Cossiga ha dichiarato più volte

siate poi conseguenti su questo tema, che non sia soltanto un voto fine a sé stesso, perché credo che poi il senatore Cossiga obbligatoriamente dovrà tornare in Aula a ripetere sempre le stesse cose, che tra l'altro io condivido.

nel rispetto delle precise norme della Costituzione, mi sembra doveroso concludere, anche a nome del Gruppo Per le Autonomie, che le dimissioni del senatore a vita Cossiga devono essere respinte. Oltre a questo motivo giuridico, vorrei aggiungere anche un motivo politico, che è quello che mi dà l'occasione per esprimere al senatore Cossiga la nostra stima per il suo operato in tutta la sua vita politica che ormai è di quasi 50 anni, per il suo operato parlamentare, per il suo operato come Presidente della Repubblica e come Presidente di questa Assemblea. Nell'esprimere questa stima, vorrei anche aggiungere la stima per tutti i senatori a vita presenti in quest'Aula, che hanno, secondo la Carta fondamentale della Repubblica, il diritto e il dovere di espletare il loro mandato secondo quanto è previsto dalla Carta stessa, con pieni diritti e doveri. Ritengo che i motivi che il senatore Cossiga ha indicato nella sua lettera di dimissioni e che ha diramato a tutti nella sua motivazione orale qui in Aula debbano dare, però, Per quanto riguarda il diritto di voto che lui mette in discussione nella sua argomentazione, non è questa la sede per decidere; noi non ci precludiamo ad una discussione generale sulla

a vita voti, commentare quel voto con giudizi politici che non hanno niente a che fare con la nostra Assemblea. Finché la Costituzione è questa, come è questa la legge elettorale che è di rango molto minore,

Per quanto riguarda, invece, l'argomentazione delineata dal senatore Cossiga, relativa alla non risposta ad

deve pertanto avere conseguenze chiare sia negli atti del Governo sia in quelli della Presidenza che ha l'obbligo di sollecitare le risposte. In conclusione vorrei aggiungere, oltre al ringraziamento parlamentare del nostro Gruppo, un caloroso ringraziamento anche da parte proprio dell'Alto Adige-*Südtirol*

mi sento in qualche misura costretto per la seconda volta - l'ho fatto nel corso della precedente legislatura - a sostenere una tesi che non è quella prevalsa in Senato nella scorsa legislatura e ritengo che non prevarrà neanche questa sera. Non parlo in dissenso dal mio Gruppo. Il collega Buttiglione ha indicato le ragioni per le quali suggerisce ai senatori dell'UDC di votare contro le dimissioni del presidente Cossiga. penso che il Senato non debba pronunciarsi in questo caso, perché ritengo che i Presidenti della Repubblica, a differenza dagli altri senatori a vita nominati dai Presidenti della Repubblica, possano soltanto rinunciare

La mia opinione, in un certo senso, tende ad accentuare al massimo il significato che la Costituzione attribuisce alla partecipazione ai lavori del Senato di chi è stato Capo dello Stato;

questa opinione nel diritto costituzionale. Personalmente, ritengo che questa sia l'opinione prevalente e da preferire. Mi rendo conto che il Presidente del Senato, mettendo all'ordine del giorno le dimissioni del presidente Cossiga, non ha opinato in questo senso non me ne rammarico: la mia era, e rimane, una personale opinione di ordine costituzionale e politico. Affermo ciò perché il presidente Cossiga, nella sua lettera, esordisce parlando di dimissioni da senatore, istituto che, secondo me, non si applica a chi ha ricoperto la carica di Capo dello Stato, e termina chiedendo al Senato di valutare le sue motivazioni e decidere sulle sue dimissioni. Come abbiamo ascoltato nei vari interventi, la valutazione sulle sue dimissioni è stata molto diversa da collega a collega e ciò non mi meraviglia. Vi è stato più un giudizio politico sul significato delle dimissioni e sulla persona che si dimette; non mi meraviglio di questo, ma, nel caso di ex Presidenti della Repubblica, lo ritengo assolutamente improprio, inidoneo e costituzionalmente non corretto. Per queste ragioni, non parteciperò al voto, perché credo che molti colleghi sappiano che ho maturato e maturo molteplici rapporti personali di grande deferenza, stima e amicizia nei confronti del senatore Cossiga, che confermo, ma che non mi fanno velo (come non mi hanno mai fatto velo) nei confronti dello stesso presidente Cossiga in materia di interpretazione della Costituzione. Per queste ragioni, signor Presidente, il mio non è un dissenso dall'indicazione del voto contrario alle dimissioni dato dal collega Buttiglione, bensì un'opinione che il Presidente del Senato,

ritenendo che lo *status* del senatore Cossiga sia indisponibile per lo stesso senatore, così come sono indisponibili una serie di diritti dei parlamentari. Vorrei fare un esempio.

Io stesso, per l'esame dei tabulati telefonici, in seguito a minacce ricevute, ho dovuto attendere l'autorizzazione a procedere da parte del Senato, perché non era un mio diritto disponibile. Parimenti, ritengo indisponibile lo *status* del senatore a vita, che lo è di diritto, in quanto è stato Presidente della Repubblica. Quindi, confermando il rapporto di

ha affrontato un problema come questo due o tre anni fa, con un dibattito che ho letto, e ha posto un punto fermo sul problema,

indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni voteranno sì, premendo il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari voteranno no, premendo il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi voteranno di conseguenza, premendo il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

dello stesso Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato (cioè 162 voti). Nella seduta di martedì 30 gennaio 2007, dopo la relazione del relatore Caruso, ha avuto luogo la discussione generale ed è stato quindi illustrato l'emendamento 1.1, a firma del senatore Stiffoni ed altri, sul quale il relatore ha espresso l'invito al ritiro; qualora non fosse ritirato, il parere sarebbe contrario. Si sono, quindi, concluse le dichiarazioni di voto sul predetto emendamento, nonché sui documenti II, nn. 5 e 6, che avevano posto il problema.

Ricordo che anche per l'approvazione di tale proposta emendativa, volta a sostituire integralmente l'articolo 5 del Regolamento, occorrerà la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. ***Votazione nominale

concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa

sarei disponibile a ritirare l'emendamento 1.102. Con una norma di legge stabiliamo un obbligo per il Governo che, attraverso un ordine del giorno, rischierebbe di essere vanificato. Credo che, proprio a tutela del Governo, che ha detto che non c'entra niente in questa vicenda, si possa sapere, di qui a due mesi, che cosa è accaduto veramente.

precedenti di norme formulate in questi termini. Dal momento che credo che sia interesse di tutto il Senato e del Governo medesimo avere un chiarimento su questo punto, voterò a favore dell'emendamento 1.101. Credo che tutta la maggioranza possa tranquillamente farlo e credo a questo punto che il Governo possa anche riconsiderare la propria posizione rispetto alla richiesta di ritiro. Naturalmente, ribadisco la contrarietà all'emendamento

«lo accogliamo come raccomandazione, se diventa ordine del giorno». Altra cosa ha sostenuto il senatore Salvi.

comprensione. Ho avuto l'impressione che il Sottosegretario volesse ripercorrere la strada propostaci degli ordini del giorno. È un'altra cosa. Stiamo parlando dell'emendamento. C'è una disponibilità;

che mira a significare che la responsabilità di aver scritto il maxiemendamento alla finanziaria non è politica, di colui che ha firmato l'emendamento, ma di un oscuro funzionario

Non ci si può nascondere dietro una foglia di fico.

colleghi, non vi siete resi conto esattamente di cosa sarebbe accaduto se l'emendamento fosse stato approvato, come spero accada invece per questo:

infatti, non può essersi autocostruito; non esiste un programma informatico che autocostruisca emendamenti. È chiaro che questo emendamento è stato pensato da qualcuno del Governo ha ordinato a qualche funzionario di introdurlo nel testo e quindi esisteva una responsabilità precisa. È del tutto ovvio, senatore Vegas, che la responsabilità politica è del firmatario del maxiemendamento, ma così facendo sarebbero emerse anche

schieramento politico - sapessero a favore di chi è stata pensata, ipotizzata, bocciata, ma poi riproposta, una norma che certamente avrebbe sancito la loro assoluta impunità attraverso

se non si vogliono applicare due pesi e due misure, per quanto possa essere difficile. Sono però sicuro che i potenti mezzi del Governo, che hanno la capacità anche di raccordare le varie procedure e di raccogliere i relativi dati, possono consentire questo *screening*.

dunque che questo emendamento possa fare chiarezza, possa far cadere tanti dubbi e possa consentire al Governo di chiarire le ragioni di questi inserimenti inopinati,

della pura necessità di fare in modo che vi siano procedure e tempi di prescrizione più rapidi, affinché il cittadino non sia sottoposto

Signor Presidente, noi del Gruppo dell'UDC non abbiamo votato a favore del precedente emendamento del senatore Storace perché non andiamo in cerca di capri espiatori non pensiamo che un oscuro funzionario debba portare la pena di un atto politico che è responsabilità complessiva di tutto il Governo.

Posso attestare che la 7a Commissione ha compiuto un bel lavoro: abbiamo lavorato bene - maggioranza ed opposizione insieme - e abbiamo approvato importanti emendamenti con il consenso dei Ministri. Tutto però è saltato, perché il maxiemendamento non ha tenuto affatto conto di quel lavoro.

Voteremo invece a favore dell'emendamento 1.102 del senatore Storace, anche se devo dire che la mia curiosità non è quella di sapere

malefatte passate. Non so quanto noi, amici dell' opposizione e della maggioranza, siamo consapevoli di un modo di agire di questo Governo che genera posizioni giuridiche future, che avrebbero assai bisogno della copertura offerta dall'emendamento Fuda. Siamo consapevoli del fatto che questo Governo si pone in Europa in condizioni che rendono prossima

e arriveranno - posizioni di condanna per il comportamento tenuto in quell'occasione, in cui siamo riusciti a metterci dalla parte torto pur avendo originariamente ragione, nasceranno responsabilità portata a carico dell'intero Consiglio dei ministri che ha approvato a suo tempo quel provvedimento. Cosa dire dei tanti provvedimenti annullati

Cosa dire di tante promozioni arbitrarie che hanno scavalcato personale della pubblica amministrazione? Cosa dire di tante sostituzioni arbitrarie all'interno di consigli di amministrazione dipendenti dalla pubblica amministrazione? Badate, l'emendamento Fuda sembra essere coerente con un progetto che mira a liberarsi dai limiti che la legge impone al potere politico. Non so quanti di voi hanno visto di recente il documento messo in circolazione sul tema della pubblica amministrazione, dei suoi diritti e dello scempio che ne viene fatto in questa fase,

com'è accaduto nel precedente emendamento. Infatti, lì non c'erano scritte le parole "un oscuro funzionario", si parlava di responsabilità; però, collega Castelli, bisogna apprezzare la libertà che c'è all'interno di una coalizione. Ne faremo tesoro per il futuro, quando esamineremo altri provvedimenti e ciascuno di noi potrà comportarsi con la stessa libertà con cui ci si è espressi in questa particolare particolare discussione. Credo che si tratta di fare passi in avanti in materia di trasparenza delle norme, per consentire ai cittadini che nessuno possa ritenersi salvo rispetto ad autentici pasticci che erano stati combinati dal Governo. La maggioranza, del resto, ha la garanzia che l'opposizione è capace di fare capriole anche su queste questioni. Resta in me grande amarezza. Spero che almeno quest'emendamento possa essere

Credo che sia interesse di tutto il Parlamento capire come sia stato possibile che una certa norma sia stata inserita e poi espunta per metà nel maxiemendamento che è stato preannunciato. La norma giuridica non c'è. Il rappresentante del Governo ha detto, tuttavia, che sarebbe stato disposto ad accogliere un ordine del giorno. Insisto nella richiesta proprio per evitare che su oscuri o meno oscuri funzionari facciano ricadere responsabilità non proprie e perché credo che il Parlamento abbia il diritto di sapere con esattezza chi ha introdotto ‑ certamente non un parlamentare, perché il maxiemendamento è del Governo ‑ quella norma.

annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 1.102 per una ragione molto semplice. Ho sempre avuto in avversione l'idea di giustizia che si basa sul tipo di autore e che fa liste di proscrizione precedenti o anticipate. Nella scorsa legislatura, l'attuale maggioranza ha inscenato per anni un'insopportabile gazzarra contro la legge e il diritto, accusando la nostra parte politica di produrre leggi *ad* *personam*, quando le leggi erano a favore del diritto, del ristabilimento della civiltà giuridica e del ripristino di uno stato di diritto che in Italia manca. Una lista di proscrizione anticipata su chi avrebbe potuto beneficiare di una norma che in questo ramo del Parlamento ci si appresta ad abrogare mi pare violi questi princìpi che nella scorsa legislatura tutto questo schieramento che oggi sembra voler introdurre tale norma aveva difeso. E mi stupisco che il senatore Castelli, che è stato esemplare nel suo ruolo di Ministro della giustizia, oggi cada in questa trappola antiliberale e antigarantista che gli emendamenti al nostro

la responsabilità di quella norma ricade in primo luogo sul presidente del Consiglio Romano Prodi ed è su di lui che devono appuntarsi tutti gli strali, compreso il suo, di questo decreto con cui si è smentito. Non si possono recitare due parti in commedia e consentire a nessuno l'alibi dell'errore materiale che è la vera vergogna del decreto in esame con cui si giustifica un atto che era politicamente cosciente

2007», con riferimento all'entrata in vigore. Per avere questa risposta, però, il procedimento contabile dovrebbe arrivare a definizione, essendo possibile la sentenza e anche l'assoluzione.

Presidente, Forza Italia voterà contro questo ordine del giorno e non per il merito, ma per la procedura che sottende. Sarebbe estremamente pericoloso pensare che una responsabilità politica - perché tale è la responsabilità da parte dell'organo proponente, il Governo, o da parte di componente del Parlamento su una norma, qualunque essa sia - potesse comportare un'attività di indagine di un ufficio giudiziario. Guardate: sarebbe un *vulnus* gravissimo. E qual è reato? E l'Avvocatura dello Stato cosa dovrebbe fare, costituirsi parte civile? E il reato quale sarebbe? Di favoreggiamento? E se domani il Parlamento o il Governo decidessero di depenalizzare un reato, ci sarebbe forse favoreggiamento di coloro che in quel momento sono indagati? Qui si rischia di mettersi sotto tutela dell'ordine giudiziario, dimenticando la libertà di opinione e di indirizzare il percorso legislativo, come meglio ritiene il Parlamento, espressione in una democrazia della sovranità popolare. Al di là delle eventuali responsabilità di carattere politico - perché non ci sono certamente responsabilità da parte del funzionario di turno - non è assolutamente pensabile che una segnalazione - certamente dispiace che la segnalazione venga da un ex magistrato, ma certamente l'ex qui è veramente più pesante del solito significato, e d'altra parte la discutibilità di tanti comportamenti in una certa stagione della nostra Repubblica danno conto della caratura anche tecnica e della voglia di giustizialismo e di controllo della libertà di opinione e della libertà di regolare legislativamente, che non può assolutamente essere negata né al Governo come espressione di una maggioranza parlamentare e come indirizzo politico e legislativo neppure al Parlamento. Allora, è fin troppo evidente e addirittura credo neppure ammissibile un emendamento, ma addirittura un ordine del giorno, ai fini della sua trasformazione in raccomandazione. si ritenesse ammissibile, non possiamo che votare contro perché metteremmo sotto tutela giurisdizionale ad ogni piè sospinto la massima espressione di una democrazia.

mi sembra che il senatore Centaro abbia espresso in maniera cristallina anche il mio pensiero. Credo che questo tra l'altro sia un ordine del giorno che presenti un *fumus* di incostituzionalità. Vi è un problema tra Parlamento e Governo e noi investiamo di questo problema un terzo potere dello Stato, qual è la magistratura, violando, secondo me in maniera patente, il principio di separazione dei poteri. Esiste uno strumento previsto dalle leggi, dai Regolamenti, dalla Costituzione, che è il potere ispettivo del Parlamento sul Governo. È il Parlamento che, caso mai, deve vedere e sindacare qual è l'operato del Governo. Questa è la prima considerazione. La seconda è che in questo momento, in cui la politica è particolarmente debole e si assiste ormai da anni ad un tentativo di invasione di campo da parte di altri poteri, sostanzialmente della magistratura di ogni tipo, per quel che riguarda l'attività politica ed amministrativa del Paese credo non sia possibile da parte nostra accettare che *motu proprio* il Parlamento o il Governo vadano in questa direzione. Credo si debba andare nella direzione esattamente opposta. Pregherei pertanto caldamente il senatore Storace di ritirare

Voglio semplicemente far notare una cosa. Se le cose che qui sono state dette hanno una coerenza, a me meraviglia la posizione che il Governo aveva assunto rispetto ad un ordine del giorno che è di natura politica, non certo giuridica, che lei si era detto disponibile ad accogliere come raccomandazione. Già questo fa capire a che livello di assurdità siamo arrivati, perché vorrei che il Governo rispondesse ai colleghi dicendo: "Ma che cosa state dicendo? Questa cosa si poteva fare". Di più, qual è il tema che ho voluto sollevare con questo ordine del giorno? Ha infatti ragione Castelli, la politica è debole, non possiamo andare ancora una volta sotto altri poteri. Ma qui è un Ministro del Governo che ha detto di rivolgersi alla procura della Repubblica di Roma contro il suo Governo. Questa è il fatto ridicolo che questo ordine del giorno denuncia. Vorrei che il Governo ci dicesse se ha ragione o ha torto il ministro Di Pietro a rivolgersi alla procura della Repubblica, quando ci scodellate un maxiemendamento su cui mettete la fiducia dicendo che non vi siete accorti della norma chiamata «comma Fuda». Credo che questa sia la valutazione politica, altro che sofismi di carattere giuridico. Lo dico anche ai colleghi che si sono intrattenuti con particolare dovizia di argomentazioni giuridiche e sono gli stessi che quando il ministro Di Pietro si rivolse alla procura della Repubblica

non vorrei mettere in imbarazzo un Gruppo parlamentare e pertanto lo ritiro.

Presidente, penso che questa sia una questione cruciale, cioè entriamo nel problema fondamentale che è stato

è possibile che la Corte dei conti possa portare avanti procedimenti *sine* *die*? È possibile che una volta che il procuratore ha attivato il procedimento per responsabilità contabile per danno erariale non vi sia più alcuna prescrizione e un amministratore che cade sotto questa mannaia non sa non sa per anni e anni se è colpevole o innocente? È possibile che tutto ciò addirittura possa ricadere sugli eredi? Credo che dobbiamo mettere un termine. Dobbiamo introdurre una prescrizione su questo tema. Ora, posso capire che entrare così, *ex* *abrupto,* su articoli del codice civile possa portare una qualche difficoltà

a colpi di emendamenti approvati a tambur battente, perché effettivamente qui si tratta non tanto di andare a toccare una norma che riguarda esclusivamente la Corte dei conti ma che riguarda il codice civile. È un'obiezione che mi sento di accettare. A questo proposito, ho già presentato all'Assemblea e alla Presidenza un ordine del giorno che andrebbe a sostituire e farebbe cadere questi emendamenti. Vorrei, però, che il relatore ed il Governo mi ascoltassero attentamente, non vorrei che quest'ordine del giorno fosse della serie «un ordine del giorno non si nega a nessuno», gradirei un impegno solenne, solenne, e che resti agli atti, da parte del Governo e del relatore, che questa materia venga affrontata quanto prima, perché questa, colleghi, è l'unica strada maestra che abbiamo di fronte: legiferare alla luce del sole, legiferare in quest'Aula su un tema che sta facendo troppe vittime, sul quale la Corte dei conti,

al collega Buttiglione: non s'illuda, collega, che la sinistra si sia costruita una norma a futura memoria, perché vede, e cito due casi: il primo è il caso Bassolino, in cui la Corte dei Conti non è mai intervenuta sulla vicenda dei rifiuti, eppure ci sarebbe materia di danno erariale sotto ogni punto di vista, questo per dire che la sinistra non teme l'intervento della magistratura, né contabile, né ordinaria. Cito poi un altro caso che credo i colleghi debbano conoscere: lo Stato lo Stato italiano paga ormai circa 250 milioni all'anno per risarcire i cittadini colpiti da sentenze troppo lunghe, interviene la legge Pinto.

altre volte vengono emesse tardi (è un caso che c'è anche oggi sui giornali) perché il magistrato competente ha, per esempio, pronunciato la motivazione con due anni di ritardo.

su questo tema. Trasformo quindi volentieri i miei emendamenti in ordine del giorno, a patto che il Governo si impegni seriamente; qui c'è il sottosegretario Scotti, per cui nutro

che toccavano il problema della disciplina della prescrizione con un allungamento dei tempi e presenta un ordine del giorno, di cui ha sottolineato il significato. Lo leggo, perché non credo sia stato distribuito. altresì i pubblici amministratori, negli eventuali giudizi a loro carico, hanno il diritto inalienabile ad un pronunciamento in tempi ragionevolmente brevi, inoltre la giurisprudenza della Corte è di fondamentale importanza per un corretto svolgimento dell'azione amministrativa, impegna il Governo: a predisporre, in tempi brevi, nuove norme

risulta agli atti, contro i suoi emendamenti in quanto consideravo sbagliato affrontare il problema dalla coda, cioè guardando al punto della prescrizione senza considerare più complessivamente il tema e soprattutto toccando istituti delicatissimi come è quello della interruzione della prescrizione. Certamente non potremmo ora, in sede di emendamento ad un decreto-legge, affrontare compiutamente il tema.

«impegna il Governo a predisporre nuove norme che tendano a tempi più brevi per l'accertamento delle responsabilità degli amministratori e il giudizio davanti alla Corte dei conti, riconsiderando in questo quadro anche i profili concernenti la prescrizione dei procedimenti».

Presidente, lei sarà sicuramente informato dell'episodio che ha riguardato una collega, cioè delle minacce ricevute, via *web*, dalla nostra collega Franca Rame che, per la verità,

Avremmo anche potuto dare un contributo maggiore, magari approvando alcuni degli emendamenti che pensavamo fossero maggiormente sostenuti. Abbiamo dato il nostro contributo per tentare un'opera di chiarificazione. un aborto giuridico non fa parte del nostro patrimonio giuridico grazie a un intervento tempestivo del Governo. Restano dei punti da chiarire. Speriamo che in seguito capiremo bene, a tutela soprattutto dei senatori che devono essere messi in condizione di svolgere sempre e comunque con serenità la loro attività, quale è stata la forza, l'energia o l'istituto che successivamente a quanto deciso in quest'Aula e in Commissione bilancio ha modificato una decisione adottata nelle sedi competenti. Concludo confermando il voto favorevole dei senatori dell'Italia dei Valori. Signor Presidente, colleghi senatori, con la votazione odierna convertiamo questo decreto integrativo della finanziaria per evitare che la norma contenuta al comma 1343 produca i suoi effetti. Già il Quirinale, subito dopo la controfirma del decreto, precisava che "La norma abrogata non sarebbe entrata in vigore con la legge finanziaria, evitando in tal modo qualsiasi ipotesi di danno per l'erario." Si è provveduto, dunque, a correggere con tempestività quello che è stato definito un mero errore redazionale, per sedare la *bagarre* di quei confusi giorni all'indomani del voto di fiducia sulla legge finanziaria. Purtroppo la discussione in Parlamento si riapre ancora per cercare un capro espiatorio, in un clima non troppo mutato rispetto a qualche mese fa che già qualcuno ha provveduto a definire di strano giustizialismo. Viceversa, penso si debba procedere con cautela non trascurando il fatto che alla base della confusione legislativa vi è un errore di interpretazione. Ritengo di non poter essere critico quindi e di condannare fermamente *escamotage* o vie di fuga non è un gioco di parole, dico di fuga, non di Fuda, che non c'entra, e che permetterebbero di incrementare l'evasione a danno dell'erario, ma al contempo flessibile nel giudicare il comma 1343. Tale posizione deriva dalla convinzione che, se l'emendamento non fosse stato estrapolato dal suo contesto originario, forse diversa sarebbe stata l'interpretazione, tant'è che lo stesso senatore ha tenuto a relazionarci, chiarendo la duplice motivazione della norma che sanciva l'effettività del termine di prescrizione e rafforzava la personalità della responsabilità nell'ambito degli illeciti legislativi. A questo punto, date le molteplici questioni politiche e tecniche che si sono innestate sul caso, questo è il momento della chiarezza, e Fuda ha cominciato a fare chiarezza. Da un lato, è assolutamente corretta la denuncia della Corte dei conti, laddove si evidenzia come una prescrizione breve della responsabilità per gli illeciti contabili, avrebbe fatto sfumare una lunga serie di cause per il risarcimento danni all'erario, con grave nocumento per il recupero di risorse finanziarie. in una logica di efficienza della pubblica amministrazione e di certezza delle responsabilità di pubblici amministratori - altrettanto corretto è il ragionamento per cui il comma in questione altro non fa se non modificare il *dies a quo* della prescrizione, anticipandolo al momento in cui si realizza la condotta produttiva del danno. Alla luce di tali valutazioni, mi chiedo se al di là delle improduttive strumentalizzazioni politiche di cui il Paese è saturo - si sarebbe potuto aprire, nella giusta sede, un dibattito approfondito sui contenuti del comma, anche se la ristrettezza dei tempi e la paventata possibilità di finire ad una gestione provvisoria del bilancio erano certamente incombenti. Da qui vorrei prendere spunto per una brevissima riflessione circa la necessità di rivedere, il prima possibile, le regole che disciplinano la sessione di bilancio. È fondamentale intervenire, così come la mia proposta di legge si prefigge, puntando ad una ridefinizione della struttura e nei contenuti e nelle procedure della manovra finanziaria di fine anno. Occorre superare, una volta per tutte, i limiti e le criticità della legge finanziaria, che si traduce oggi in un complesso di disposizioni di portata sempre più ampia ed eterogenea, coacervo di norme della più varia natura, che risulta difficile, per non dire impossibile, analizzare e approfondire come si dovrebbe: forse, in tal modo, inconvenienti come quello creato dal cosiddetto emendamento Fuda difficilmente potrebbero sorgere. In conclusione, a nome del Gruppo Popolari-Udeur, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di conversione. *(Applausi

troviamo qui a discutere su un ennesimo tentativo del Governo in carica di porre rimedio ad un proprio vistoso errore: questo, perlomeno, è conclamato. Certo, questa volta Prodi si è venuto a trovare - come si suol dire - tra l'incudine e il martello: pressato dalla propria traballante maggioranza; smascherato da un'opposizione consapevole del proprio ruolo; in evidente difficoltà per dover trovare una giustificazione plausibile a quello che si è voluto far passare come un mero errore tecnico, cerca ora, in quest'Aula, con questo disegno di legge, di mettere a tacere la polemica sorta intorno al comma 1343 dell'articolo 1 Un comma fantasma, oserei dire, senza genitori o con doti di prestigiatore: comparso dal nulla dopo essere stato bloccato dal Governo stesso e dalla sua maggioranza, riscompare oggi o, forse, è questo che vogliono farci credere; un comma nascosto, occultato nell'ambito di una caotica e disordinata manovra, comunque sconosciuta ai suoi stessi sostenitori, che, per non rischiare le proprie poltrone, hanno approvato un provvedimento finanziario alla cieca. Il gioco, però, evidentemente non è ben riuscito e i cosiddetti indipendenti presenti nel Governo non hanno esitato a lavare i panni sporchi in pubblico. Di certo, non posso dire di avere invidiato la posizione di Prodi, ma non sarebbe la prima volta: si può forse pensare che ormai vi abbia fatto l'abitudine. sappiamo bene che, in realtà, di un errore non può essersi trattato: la verità è anche mal simulata. Non era necessario il biasimo della Corte dei conti, che denuncia, nel caso in cui non si intervenga, l'estinzione di almeno il 60 per cento dei procedimenti in corso, grazie all'applicazione del principio del *favor rei*; sarebbe, forse, interessante poter verificare in concreto, invece, i nomi di molti degli amministratori coinvolti da tale sanatoria

Non vogliamo buttarci in una forsennata caccia alle streghe: a questo ci ha già pensato un Ministro di prestigio (anche dal punto di vista giuridico); senza esito, tuttavia, visto che il senatore Fuda ha rigettato - e credo a favore - qualsiasi colpa. però, al punto e abbandonando il sano sarcasmo che ci contraddistingue, la questione - annosa e complessa - merita sicuramente un intervento più attento nell'ambito di una globale rivisitazione del sistema giustizia (recupero, pertanto, gli interventi del senatore Castelli

voteremo in senso contrario al provvedimento in esame, in segno di protesta all'agire complessivo di questo Governo e soprattutto per ribadire la nostra posizione fortemente contraria all'intera manovra finanziaria. Voteremo in senso contrario, perché non è possibile per un Governo degno di questo nome agire in questo modo, ledendo la credibilità dell'intero sistema. Una norma come quella oggi in discussione, produttiva di effetti così palesemente *ad personam*, il tentativo di farla passare per un errore, ci sembra un maldestro espediente per offuscare l'opinione pubblica. Il gioco non è riuscito e si arriva oggi qui, tentando di coinvolgere anche il Parlamento in questa semifarsa. Noi allora ne approfittiamo anche per chiedere, anzi per pretendere, che finalmente questo Governo si impegni in qualcosa di realmente serio e pensiamo ad una riforma della giustizia. Infatti, se le parole del ministro Mastella dell'altro giorno fossero applicate e i tempi della giustizia fossero davvero dimezzati, potremmo anche non chiedere provvedimenti come quelli di Fuda, perché sarebbero inutili, visto che le lungaggini dei tribunali dovrebbero essere essere un'esperienza del passato. Chiediamo una riforma del procedimento di formazione della legge finanziaria, come del resto anche la maggioranza stessa e il ministro Chiti hanno chiesto più volte, che impedisca di renderla una legge *omnibus*, in cui inserire a tradimento tutto ciò che si ha interesse a far approvare. Pretendiamo un Governo all'altezza del suo compito, ma forse, per questa legislatura, pretendiamo un po' troppo.

per effetto dell'inserimento nel maxiemendamento al disegno di legge finanziaria per il 2007 di una modifica alla legge n. 20 del 1994, i termini di prescrizione per la perseguibilità dell'illecito contabile sarebbero stati collegati alla realizzazione della condotta produttrice del danno erariale e non al momento della verifica della lesione stessa, come invece previsto dalla disciplina attualmente in vigore. La retrodatazione del giorno dal quale iniziare a far decorrere i termini della prescrizione contabile, avrebbe avuto come probabile effetto, da una parte, una generale amnistia per la pratica difficoltà di individuare il momento in cui la condotta è posta in essere e per il raggiungimento dei cinque anni di tempo a disposizione della Procura contabile in maniera molto più facile dell'attuale e, dall'altro, la conduzione in giudizio di casi destinati al proscioglimento per assenza del danno erariale. Sostanzialmente, negli illeciti contabili perseguibili per danno erariale, la prescrizione sarebbe scattata prima ancora che il danno si fosse compiuto: una prescrizione super anticipata, è stata definita, un colpo di spugna, come denunciato dal Procuratore generale della Corte dei conti, che rischiava di vanificare il recupero di 310 milioni di euro per illeciti contributi agricoli dell'Unione Europea e così per le consulenze d'oro, per la responsabilità di amministratori di società a capitale misto o partecipato, dall'Alitalia, all'ENEL, alle aziende comunali. Con l'ulteriore risultato collaterale di creare probabilmente un mostro costituzionale. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non si può far decorrere la prescrizione di un'azione che non si può ancora esercitare perché non è verificato il danno erariale. Ricordo che un ulteriore duro allarme era arrivato anche dall'Alto Commissario anticorruzione che, in una nota, aveva denunciato il rischio di chiusura dell'organismo che presiede, in caso di entrata in vigore di questo emendamento. Dalla maggioranza sono arrivati segnali immediati della volontà di cambiare la norma, ma al Senato, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione prima del voto di fiducia e l'assenza, va ricordato, di un unanime consenso verificato dal presidente Marini, tre le forze politiche dell'opposizione, modo, impraticabile è stata la possibilità di un intervento della Camera che avrebbe obbligato l'intero provvedimento ad un ritorno a Palazzo Madama, con il rischio dell'esercizio provvisorio. Pertanto, nel rispetto degli impegni assunti al riguardo, con la sua maggioranza, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con assoluta tempestività sul testo della legge finanziaria per per evitare che la predetta disposizione potesse cominciare a produrre effetti nel sistema normativo vigente, e lo ha fatto con il decreto-legge che è sottoposto alla conversione da parte di questa Camera. è stato affermato che l'inserimento di questa norma è risultato il frutto di un mero errore redazionale. Qualcuno su questo ha sorriso, qualcuno ha ironizzato, qualcuno ha cercato i colpevoli. Tuttavia va detto - ed è un dato di fatto - che l'eccezionale complessità della legge finanziaria, in particolare quella per il 2007, composta da quasi 1.400 commi, se non è la la causa che ha determinato l'introduzione in quel provvedimento di una norma, appunto il comma 1.343, censurabile sia nella sostanza sia nella sede in cui è stata disciplinata la materia,

che quest'Aula abbia approvato con la fiducia un maxiemendamento che conteneva anche questa norma. Poiché le regole spetta a questo Parlamento farle, credo che in questo caso vada ribadita l'esigenza di introdurre regole nuove e procedure parlamentari che consentano effettivamente a tutti noi di valutare con piena consapevolezza e trasparenza quali sono le proposte che sono sottoposte al voto. È nostra responsabilità, infatti, non tanto e solo cercare la manina - com'è stata definita - che ha inserito questo comma, ma mettere in condizione l'Aula che questo non si ripeta. Se le regole sono chiare e trasparenti, il rischio che questo accada di nuovo e la necessità di cercare fantomatici colpevoli sicuramente saranno minori. Il problema della prescrizione degli illeciti contabili è problema annoso. Ricordo che tali illeciti erano considerati imprescrittibili. La prescrizione fu poi stabilita in dieci anni. Nel 1996 è stata ulteriormente ridotta a cinque anni, con esplicita esclusione degli eredi, salvo che in caso di ingiusto arricchimento. una decisione ineccepibile, perché non è ragionevole sottoporre gli amministratori pubblici al rischio di richieste contabili eccessivamente protratto nel tempo e destinato addirittura a trasmettersi agli eredi in caso di morte. Ciononostante, in un Paese in cui i malanni della giustizia sono noti, gli amministratori continuano a vivere con angoscia l'incombenza della giustizia contabile che opera, giustamente, con grande severità sulla base di prassi rigoristiche, subordinando la condanna non al dolo, ma alla semplice colpa dell'amministratore, determinando sovente obblighi di pagamento all'erario molto elevati. Bisogna anche dire che taluno rischia di essere perseguitato, sempre per i famosi malanni della giustizia nel nostro Paese, altri ingiustamente non sono affatto incriminati e perseguitati. Non di meno, indebolire indiscriminatamente la giustizia contabile sarebbe pericoloso, poiché in assenza di un controllo giurisdizionale adeguato si rischierebbe di incentivare una gestione del denaro pubblico caratterizzata da sprechi senza freno in un Paese, come il nostro, dove lo spreco del pubblico denaro costituisce purtroppo una piaga diffusa. Per questo motivo la difesa d'ufficio delle ragioni degli amministratori pubblici scialacquoni, da chiunque provenga, non è condivisibile. Certo, nessuno può essere considerato reo a vita. Tuttavia, già oggi in Italia, nessuno rischia in realtà condanne per illeciti imprescrittibili. Occorre, dunque, evitare - e lo facciamo con il voto di oggi - che attraverso una modifica surrettizia delle regole della prescrizione degli illeciti contabili centinaia di procedimenti rischino - come ha denunciato la Corte dei conti - di estinguersi con danni incalcolabili per l'erario. In questo senso il Governo, su forte e pressante indicazione di questa maggioranza, ha operato giustamente con tempestività per rimediare all'indebito inserimento dell'emendamento in questione in finanziaria, perché l'interesse ad una gestione irreprensibile della cosa pubblica deve comunque prevalere su tutto. L'attenuazione dell'incisività dei controlli, anche soltanto attraverso la modificazione delle regole della prescrizione, invece di aprire la via ad un'illegalità ancora più devastante di quella che ha già sufficientemente colpito fino ad oggi il nostro Paese. Le istituzioni più alte del Paese, tra cui quest'Aula, hanno il dovere d'affermare che se ogni illegalità è inaccettabile, tanto più inaccettabile è se si tratta di illegalità commessa da chi è investito di pubbliche funzioni. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

e io non ho difficoltà ad affermare che il Governo è scivolato sulla classica buccia di banana. È una questione che ha avuto un effetto importante sui *mass media* che, con enfasi, hanno riportato la notizia di una legge *ad personam*, che prescrive tutti gli illeciti contabili, inclusi quelli conseguenti ad accertati fatti di corruzione, di indulto contabile, di colpo di spugna degli illeciti commessi dalla classe politica e dagli amministratori locali, con conseguente impedimento da parte dello Stato di recuperare le somme delle quali funzionari e dipendenti corrotti si sono appropriati. C'erano e ci sono stati ovviamente tutti gli ingredienti dello *scoop* giornalistico: l'impunità della classe, la sottrazione delle risorse all'erario, l'indignazione della magistratura contabile, la classica sanatoria. All'opinione pubblica è arrivato un messaggio non equivoco. Noi della maggioranza, l'Unione, dopo aver avversato nella passata legislatura e combattuto

con l'aggravante del sotterfugio, di un'iniziativa poco trasparente, tradendo la fiducia degli elettori. Non abbiamo alcuna difficoltà ad affermare che

Il tema della giustizia contabile dev'essere affrontato e va posto all'attenzione del Parlamento in modo corretto, nella sede appropriata, con un esame approfondito da parte delle Aule parlamentari e non attraverso un emendamento,

per poter risolvere in modo definitivo e con tempi certi la questione al fine di punire, in tempi certi, chi commette illeciti e far incassare all'erario le somme derivanti dal risarcimento del danno. La questione dei tempi è dirimente. Si porta sempre l'esempio dei giudizi di materia espropriativa, che hanno una durata ultradecennale. Da ciò consegue che la Corte dei conti inizia l'azione di responsabilità ben oltre il termine di cinque anni. Il problema è infatti particolarmente sentito dagli amministratori

Ciò che è accaduto con la finanziaria è da ritenere un atto sconsiderato, che ha avuto come unico effetto quello di minare la credibilità della nostra maggioranza e del Governo. I problemi del Paese vanno risolti senza scorciatoie, in modo trasparente, alla luce del sole e con un esame approfondito da parte delle Aule parlamentari.

si opera con un decreto quando la finanziaria non è ancora entrata in vigore. È una soluzione già sperimentata con successo nel 2003 dal centro-destra, che abrogò per decreto una norma della finanziaria sui compensi per i dirigenti (mi ricordo che ci fu anche un richiamo da parte dell'allora presidente Ciampi) prima che la finanziaria entrasse in vigore. Per concludere, signor Presidente, vorrei

Mi riferisco, per esempio, all'errore - questo sì errore di trascrizione - relativo alla norma sulle rottamazioni senza obbligo di acquisto di una nuova autovettura, perché la norma

o veicoli di quel tipo. Tale questione mi sembra sia in via di risoluzione, poiché questa norma è stata inserita nel decreto sulle liberalizzazioni.

perché, in pratica, si bruciano negli inceneritori schifezze che producono danni all'ambiente e alla salute dei cittadini e poi si prendono degli incentivi

Tale questione non riguarda solo gli ecologisti, ma tutti coloro che sono attenti al normale funzionamento del mercato, perché vi sono aziende che agiscono

D'altra parte, era ovvio che - essendo in presenza di un errore grave dal punto di vista politico, come quello di aver inserito nel nel maxiemendamento il comma 1343 - un errore di quel tipo potesse e dovesse essere stigmatizzato aspramente dall'opposizione e dalla stessa maggioranza. Bisogna

fu chiesto di stralciare il comma 1343, proprio perché non era accettabile che un comma di quel tipo figurasse nel maxiemendamento dopo che l'argomento, trattato in sede di Commissione bilancio, era stato considerato inaccettabile. È abbastanza comprensibile che, da parte dell'opposizione e in particolare da parte di un collega come il senatore Storace, si cogliesse la palla al balzo per costruire attorno a questo

Non c'è dubbio che la questione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti e dei pubblici ufficiali sia rilevante.

Quindi, se di disattenzione si è trattato, l'invito a che il Governo sia più attento nel definire norme di questa portata è pressante. D'altra parte, il fatto che si sia parlato nella relazione di presentazione del decreto‑legge di un mero errore materiale, mi pare che dimostri con tutta evidenza come ci sia un disconoscimento totale da parte del Governo, del quale voglio prendere atto e dare atto al Governo, all'invito, appunto, a lavorare attorno alla prevenzione degli errori e non alla riparazione postuma degli errori compiuti.

interloquendo con il presidente Castelli, su un tema che a me pare di enorme rilevanza: il fatto che anche i pubblici amministratori o i pubblici dipendenti, che si siano resi responsabili di

Dobbiamo chiederci se c'è - ed io penso che ci sia - una connessione diretta tra il venir meno dei meccanismi democratici di controllo sull'amministrazione pubblica e la scelta

cioè dall'elezione diretta dei Presidenti anche delle Regioni, a partire dalla spoliazione delle funzioni di controllo da parte dei Consigli, noi abbiamo come unici riferimenti il TAR e la Corte dei conti. Vediamo quanto sia cresciuto in termini abnormi il potere del tribunale amministrativo e come ormai non ci siano più tempi certi e garantiti per i pronunciamenti. Per la Corte dei conti vale lo stesso principio. Nel ragionare come dovremmo fare e come si è impegnato a fare anche il Governo, dobbiamo essere lungimiranti e capire che dobbiamo ripristinare meccanismi e modalità di controllo interno e strumenti di controllo che attengono alla responsabilità politica e democratica degli organismi propri del nostro

contrapposizioni accese, lotte politiche, dialettica anche aspra, ma con degli avversari leali, che si

Possiamo anche capire che, dopo la figuraccia che questa maggioranza ha incamerato con l'indulto, viga la regola che è meglio usare un po' di ipocrisia piuttosto che dire veramente dove si vuole andare a parare. L'obiettivo era chiarissimo e lo ha smascherato un senatore della maggioranza: accorciare i tempi della prescrizione. Punto. Basta. Non è stato un errore. errore. Uno dei nostri colleghi, che è stato presidente di un'importante festa del cinema a Roma, potrebbe d'ora in poi organizzare il festival dell'ipocrisia perché in questa sede si è consumata una delle migliori rappresentazioni italiane. Abbiamo sentito dire

dicendo che anche la maggioranza di centro-destra ha commesso qualche piccolo pasticcio. Vivaddio! Mettiamo pure in piazza tutti questi pudori. Non si sa più come aggiustare giustificare una piccola nefandezza. Si pensa che questa norma abrogativa serva a lavarsi un po' la coscienza. Ma ormai non serve più a niente, nel senso che il nostro voto, qualsiasi esso sia, sarà irrilevante. Lo ripeto perché almeno a verbale, a futura memoria, resterà: sarà irrilevante. Per legge potremo anche scrivere che da domani il cancro si cura con l'aspirina, però, nelle facoltà di medicina, negli ospedali, i chirurghi continueranno ad asportare tessuti, i radiologi a bombardarli e se ne «fregheranno» delle sciocchezze scritte, che non hanno attinenza con la pratica, in questo caso medica. Nelle università si continuerà ad insegnare che una norma può, sì, abrogare, ma un'altra norma vigente, non una norma non ancora entrata in vigore. E dal momento in cui una norma vige, nessuno potrà scardinare il principio del *favor rei*, richiesto da chiunque sia sottoposto a giudizio, che si veda applicare la norma più favorevole, anche quella entrata in vigore per un solo minuto e poi

Penso che qualunque giudice cui ricorrerà qualunque cittadino dirà che l'urgenza e la necessità non c'erano. L'altra preoccupazione è che il provvedimento non è idoneo a raggiungere gli obiettivi che noi tutti vogliamo. Lo abbiamo detto in Commissione; abbiamo chiesto di rafforzare le motivazioni dell'urgenza e della necessità, chiedendo al Governo di presentare documentazione sul dramma e sui problemi conseguenti all'applicazione di quel comma il Governo correttamente ci ha presentato una relazione del procuratore generale della Corte dei conti, che ci ha indicato una situazione devastante, qualora questo provvedimento non dovesse passare.

nonostante tutte queste considerazioni, nonostante la linearità di posizione di Alleanza Nazionale, si è andati avanti senza muovere niente, salvo l'approvazione di alcuni ordini del giorno, che rappresentano

e non crediamo che sia scandalosa la posizione del procuratore generale della Corte dei conti che ha mandato un documento nel quale si dice che va sottolineato il rischio che l'entrata in vigore del comma 1343 vanifichi il recupero di ingenti importi, come i 32 milioni di euro versati dal Comune di Roma in esecuzione di una condanna. Ma ci rendiamo conto? Noi andiamo alla ricerca delle responsabilità e il procuratore generale già ci ha indicato una grave responsabilità e quindi un eventuale teorico interesse a quell'emendamento. Questo va detto,

però un impegno del Governo rispetto a queste nostre preoccupazioni: sia il Governo pronto a intervenire con provvedimenti d'urgenza, perché il parametro

sicuramente ci saranno ricorsi, ci sarà la giurisprudenza che dovrà dirimere questi casi e questa incertezza, che, ahimè, la disposizione determina. Con queste riserve e con questo invito al Governo di essere pronto ad intervenire, confermo il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

Signor Presidente, a nome del Gruppo UDC, come è stato anticipato in discussione generale questa mattina dal capogruppo D'Onofrio, preannunzio che voteremo a favore dell'abrogazione del comma 1343, che già abbiamo avuto modo di denunciare in sede di dichiarazione di voto alla fiducia sulla finanziaria 2007. Avevamo già in quella sede sottolineato la gravità di quanto è accaduto. Questa mattina, al di là della responsabilità di carattere individuale, il presidente D'Onofrio ha voluto insistere, e torniamo a insistere, sulla responsabilità politica. Certamente ci siamo trovati già nel passato a registrare casi analoghi, ricordo la finanziaria 2003. la finanziaria 2003. Ciò accade quando la finanziaria non ha un trasparente sviluppo in seno alla Commissione e attraverso un dibattito in Aula, ma in in stanze abbastanza riservate, a margine di quella trasparenza del dibattito politico di cui l'opinione pubblica in generale dovrebbe godere. certamente far riflettere la maggioranza sulla necessità di riformare le procedure della legge di bilancio, ma dovrebbe anche consigliare di tenere un atteggiamento diverso per favorire una maggiore trasparenza nelle sedi istituzionali in cui si forma la volontà di questo Senato e, direi, dell'intero Parlamento. Vorrei sottolineare sul punto che il merito di questa denuncia è sicuramente della maggioranza, e ricordo l'intervento molto deciso della presidente Finocchiaro in quella occasione. Diamo atto, quindi, ad una parte della maggioranza di aver posto tale questione, però non si può sottacere in questa fase che esponenti illustri, in quanto rappresentanti dei Gruppi, come ha ricordato il presidente D'Onofrio questa mattina, avevano presentato essi stessi degli emendamenti in tal senso. Quegli emendamenti, è vero, come ha ricordato il senatore Fuda questa mattina, avevano un'articolazione molto più compensativa rispetto alle responsabilità di carattere patrimoniale da parte dei pubblici dipendenti o degli incaricati di pubblici uffici. Di quei due emendamenti presentati da autorevoli rappresentanti di questa maggioranza, però, nella finanziaria è andata a finire soltanto una parte: le prime due righe, quelle due righe che hanno scardinato il buon intento, da parte di questi autorevoli rappresentanti della maggioranza, e hanno dato un risultato tutt'altro che positivo. Quindi, collega Fuda, sicuramente lei aveva dei buoni intenti, insieme ad altri autorevoli colleghi dell'Italia dei Valori, della Margherita, dei DS e quanti altri hanno sottoscritto quegli emendamenti, però certamente poi lo spirito che ne è stato portato all'attenzione del voto dell'Aula è stato tutto diverso. sapevate bene - non è stato un errore materiale - quello che volevate fare, perché siete partiti da lontano con degli emendamenti e di questi emendamenti soltanto la parte più favorevole dichiarato - di autorevoli Ministri di questo Governo. Sottolineo ancora che i beneficiari di quella norma, così come estrapolata dagli emendamenti che erano stati sul punto presentati, avrebbero beneficiato di questo accorciamento della prescrizione. Mi lego, per concludere, alle riflessioni che faceva

però una corrente dottrinaria, che si è espressa anche attraverso il dibattito sulla stampa, che ritiene invece possa applicarsi il principio del *favor rei* su questa normativa. Io spero che, in sede di applicazione della norma, il principio del*favor rei*, che non è da escludere completamente dal punto di vista del dibattito giuridico in atto, non possa rivivere, perché in questo caso tale norma avrebbe nome e cognome dei destinatari,

Le voglio dare atto che, con la sua proposta, lei poneva un problema effettivamente esistente e del quale forse sarebbe opportuno che il Senato si interessi. Le voglio, altresì, dare atto che il comma 1343 della finanziaria non ha nulla a che vedere con il suo emendamento, essendo sostanzialmente lo stralcio esclusivamente di una piccola parte, con l'omissione di tutta l'articolazione del suo progetto. A nome del Gruppo di Forza Italia, le voglio poi manifestare solidarietà per l'aggressione personale e politica di cui ella è rimasto vittima, quella solidarietà che a ben vedere non le è stata mai rappresentata dai componenti della sua maggioranza, se è vero, com'è vero, che lei è rimasto purtroppo l'unico pubblico capro espiatorio di un atto irresponsabile, esattamente quel comma 1343. Un comma che, per essere chiari, a detta del procuratore generale della Corte dei conti, avrebbe comportato l'estinzione di 3.861 procedimenti contabili con condanna in primo grado, nonché il venir meno del recupero di un importo pari a circa 4 miliardi di euro, e cioè sostanzialmente più di un decimo della finanziaria. senatore Fuda, forse abbiamo scoperto chi è il responsabile di questa operazione, nel senso che il Governo ci è venuto a comunicare che tutto si addebita ad un oscuro funzionario che, incaricato - immagino in sede politica - di espungere il suo emendamento dalla finanziaria, attraverso dei giochetti informatici per parole chiave, per parole chiave, aveva eliminato tutto quanto il suo emendamento ad eccezione del primo comma. Un'operazione, quindi, gravemente negligente da parte di un funzionario, sicuramente sciatta e questo - devo dire la verità - atteso l'omesso controllo da parte di chi, in sede politica, quella espunzione aveva chiesto, denota quantomeno quanto siano prive di fondamento quelle mielose affermazioni autoreferenziali del presidente Prodi, per cui finalmente la serietà è arrivata al Governo. Vedete, signor Presidente, signori senatori, noi riteniamo di non poter credere a quello che ci dice il Governo, non solo e non tanto per la ridicolaggine della giustificazione addotta, perché ci troviamo di fronte ad un Governo che ha come abitudine quella di modulare la verità secondo i suoi gradimenti. Un esempio per tutti: il Governo, rispondendo a un ordine del giorno presentato da un senatore dell'opposizione, ha affermato, in termini chiari, che non vi era alcun impegno da parte del Governo di centro-destra in merito all'allargamento della base di Vicenza eppure, subito dopo, per sanare le contraddizioni politiche tutte interne alle sua maggioranza, il presidente Prodi ha detto che praticamente quell'allargamento altro non era che mantenere un impegno preso dal precedente Governo. *(Applausi dal Gruppo FI*). Cosa che, alla luce di quanto detto dal Governo stesso, è falsa. Sarebbe interessante, a dire il vero, anche conoscere i nomi dei soggetti che in qualche modo avrebbero potuto beneficiare del comma 1343, ma per questo vi sarà tempo con il sindacato ispettivo. Certo è che se quella lista di nomi dovesse - come dire - presentare qualche anomalia o qualche dato di interesse, avrebbe ragione il senatore Centaro quando prima, in un suo intervento, ricordando la modifica del reato di abuso in atti d'ufficio - che tanto bene fece al presidente Prodi - ovvero quella stessa norma che si trovava nella finanziaria e che era puntata contro un illustre oncologo, sostanzialmente diceva che voi siete abituati a predicare bene, ma a razzolare molto, molto male. Avete ritenuto con un decreto-legge di dover risolvere il problema, un problema enorme, più di un decimo della finanziaria. No, senatore Bonadonna, non si è trattato di un disconoscimento (mi consenta, lo dico con molto garbo); credo si sia trattato semplicemente di una pezza a chi è stato scoperto in un tentativo molto interessato. Ebbene,

come in dottrina vi è poca materia sul punto e che sostanzialmente da parte di taluno si afferma che è possibile l'abrogazione, da parte di talaltro si afferma esattamente il contrario. Non a caso noi avevamo proposto di percorrere una strada diversa perché, nell'eventualità in cui si dovesse ritenere che l'abrogazione è possibile solo con riferimento ad una norma vigente, si avrebbe evidentemente la vita del comma 1343, sia pure per un secondo, quello utile, con buona pace del presidente Finocchiaro, per muovere tutti i meccanismi che sono propri degli istituti di diritto sostanziale. Voi continuate, avete insistito e avete dichiarato ripetutamente inammissibile il nostro emendamento e quindi si arriva alla formulazione a cui oggi si arriva. Voi stessi ritenete che forse vi è una retroattività della prescrizione: in tal senso forse lo stesso decreto-legge, in tal senso l'intervento della senatrice Rubinato; ma in tal senso, principalmente, la lettera del procuratore generale della Corte dei conti, il quale, nell'affermare ciò che ha affermato, evidentemente non ha tenuto in gran conto la giurisprudenza in base alla quale non vi è possibilità di retroattività per la prescrizione. Questo è tutto. Io credo che in questa vicenda il Governo e la maggioranza abbiano una grossa, enorme responsabilità politica. Senza fare il gioco delle tre carte, la responsabilità politica risiede nel fatto di avere inserito nella legge finanziaria un atto di grave irresponsabilità e poco importa, senatore Storace, sapere chi è il funzionario. Ciò che rileva è che il Governo, nella legge finanziaria, ha prodotto il comma 1343; ciò è ancora più grave se si pensa che quel funzionario era stato incaricato di espungerlo dal testo.

il comma 1343 entro il 23 dicembre, data di approvazione della finanziaria, e ritornare al Senato per la definitiva approvazione; ma tant'è. Probabilmente il presidente Prodi e i *leader* della maggioranza sono talmente sicuri della stabilità della loro coalizione da ritenere che in qualche modo il periodo delle festività natalizie poteva incidere sul mantenimento della maggioranza. Ma quale esercizio finanziario! La realtà è che voi avete avuto paura che quella modifica non fosse passata al Senato per l'assenza di vacanzieri del centro-sinistra. Sto terminando, signor Presidente. Vi auguro

coalizione politica, poiché avete dimostrato, ancora una volta, in questa vicenda la vostra superficialità e - se mi consentite - la vostra arroganza, ma per il Paese che davvero non merita il mancato recupero di oltre 4 miliardi, ossia più di un decimo della vostra legge finanziaria.

Il voto di Forza Italia sarà favorevole, e vorrei rispondere al senatore che mi ha interrotto. Vede, Presidente, nel dubbio dottrinario in ordine alla capacità abrogativa di una norma vigente o non vigente, Forza Italia non si vuole assumere la responsabilità, in qualsivoglia modo, di essere coinvolta in una vicenda che è nata, è vissuta e continua a vivere per mera ed esclusiva responsabilità del centro‑sinistra, di questa maggioranza e di questo Governo.

norma non venne per decisione dei Capigruppo dell'attuale opposizione. Questo è un dato di fatto che ognuno può giudicare. Certo, rimane aperta la questione del chiarimento politico con il Governo. Trovo singolare che anche qui il senatore Saporito faccia allusioni ad alte responsabilità all'interno del Governo e Forza Italia continui a parlare - non capisco il perché - di oscuri funzionari, mentre il punto è molto semplice.

Si è parlato oggi della Corte dei conti. È stato approvato anche un ordine del giorno. È giusto che il Governo si dia l'obiettivo di cinque anni per la durata di tutti i processi, non si vede perché non debba prefiggerselo anche per i processi contabili. Il problema, però, è molto più rilevante (e sono preoccupato quando i politici se lo pongono soltanto sul versante che li può riguardare) perché è di un Paese che ha smantellato responsabilità e controlli nell'agire politico.

alcuni sono stati accolti; su altri si è sbagliato e ora si rimedia; su altri sono stati commessi errori. Con altri autorevoli esponenti di tutti i Gruppi della maggioranza, abbiamo presentato oggi emendamenti per rimediare ad altri due errori che vi sono in finanziaria - chiamiamoli così - che che riguardano i tetti retributivi per i *manager* e per i dirigenti pubblici; il Presidente del Senato li ha dichiarati inammissibili. Rispetto sempre le scelte dei Presidenti del Senato,

Corte dei conti, vi è un fatto scandaloso (abbiamo proposto un emendamento in materia, che non è stato accolto): l'assicurazione che fanno gli enti pubblici dei propri amministrati per responsabilità contabile (il caso più clamoroso è quello della RAI, sulla quale sta indagando la procura della Repubblica di Roma). È giusto che un ente faccia pagare ai propri cittadini l'assicurazione per il danno subìto dai medesimi? Poniamo tali questioni perché vediamo accrescersi il rischio di sfiducia e di distacco dei cittadini nei confronti del sistema politico e delle istituzioni: anche su questo punto il Presidente della Repubblica ha proferito parole che devono essere accolte. E allora, almeno su questi temi, rifuggiamo dallo scontro, dal pretesto, dalla volontà di fare polemiche su tutto. In ogni caso, questa battaglia della maggioranza del Senato, iniziata con la legge finanziaria e che intendiamo portare avanti, ad oggi - grazie al concorso del Governo, che ha immediatamente accolto la nostra richiesta di un decreto‑legge per eliminare per eliminare questo *vulnus* presente nella legge finanziaria - è un tema più importante delle meschine polemiche su questo o su quel punto, su questa o su quell'altra questione. Per tali ragioni, esprimiamo un voto convinto a favore della conversione del decreto‑legge

Dopo tutta questa discussione, sta nascendo in me la convinzione che il colpevole, come nei migliori gialli, sia il maggiordomo, perché altri non ne ho individuati*.